affronto volentieri il tema che impegna la discussione di questi giorni, politica e non solo, dal momento che coinvolge ancor di più gli addetti ai lavori del nostro sistema economico, perché l'offerta di acquisto da parte della FIAT nei confronti della Chrysler e della Opel pone un problema di simmetria istituzionale. Infatti, mentre sia nel caso statunitense sia in quello tedesco le imprese coinvolte applicavano modelli partecipativi, l'uno in relazione alla proprietà di quote di capitale e l'altro alla presenza nel consiglio di sorveglianza di rappresentanti dei lavoratori, forme strutturate di partecipazione in Italia non esistono su base normativa, nonostante l'indicazione costituzionale dell'articolo 46. Quindi, io chiedo: qual è la valutazione del Governo sull'introduzione di meccanismi di incentivazione alla partecipazione dei lavoratori alla vita dell'impresa, con particolare riguardo alla partecipazione finanziaria? Ritiene poi il Governo che debba essere modulata una via italiana alla partecipazione, per adattarla alla speciale mappatura del nostro sistema produttivo concentrato sulle piccole e medie aziende?

e sulla loro capacità di remunerare adeguatamente le prestazioni e di garantire, ad un tempo, condizioni di accessibilità degli individui e delle famiglie alla spesa. I dati resi noti in questi giorni dall'OCSE confermano una condizione molto grave per il livello delle retribuzioni da lavoro dipendente in Italia, sia in termini di valore assoluto, sia relativamente al carico fiscale che si sviluppa nel tempo in termini inversamente proporzionali alla consistenza dei salari medesimi e che risulta tra i più pesanti nel repertorio dei 30 Paesi. I dati dell'analisi retributiva, avviata qualche tempo fa dalla Commissione lavoro del Senato, confermano, purtroppo, questa condizione che si è strutturata nel tempo, determinando negli ultimi 15 anni un appiattimento di fatto dei salari che risultano in Italia inferiori del 30 per cento a quelli medi dell'Unione europea a 15, e che sono cresciuti, negli ultimi dieci anni, sempre in termini netti, soltanto delle 0,4 per cento. Il dato è ovviamente fatto a prezzi costanti. È del tutto evidente come tale situazione non sia sostenibile, ancora più se ravvisata nel quadro della crisi attuale. Tralascio, in questa sede, le considerazioni che lei ha recentemente svolto circa le cause e le responsabilità di questa condizione, che personalmente ritengo sbagliate e volutamente mistificatorie. Colgo questa occasione per richiamare il fatto che, invece, positivamente, fra le soluzioni da lei ravvisate per affrontare queste criticità, ci sia anche il percorso parlamentare della normazione in materia di partecipazione dei lavoratori all'impresa. Su questo tema, al quale noi siamo fortemente interessati - c'è un disegno di legge a prima firma del senatore Treu, sottoscritto da tutti i senatori della 11a Commissione - abbiamo la necessità di chiarire con lei, in questa sede,

ella ritenga che in merito al rapporto tra strumenti per la partecipazione dei lavoratori alle imprese e contrattazione ai diversi livelli (nazionale, territoriale e aziendale) vi debba essere sovrapposizione e come debba intendersi l'invito, da lei rivolto ieri alla Commissione lavoro, a valutare la possibilità che i contratti aziendali di partecipazione possano, in relazione a condizioni concrete, sancire deroghe ai contratti collettivi di lavoro. Ministro, avrei due domande da porle per cui devo essere estremamente sintetico. Parliamo di dati ormai assodati: il calo dei consumi è un problema estremamente preoccupante, perché non è più solo di carattere assistenziale, ma l'erosione del potere di acquisto dei salari è diventato un problema di carattere economico. Abbiamo visto che i salariati italiani sono i meno pagati dell'area UE.

aree geografiche ha infatti dovuto fare un adeguamento standardizzato. Oggi, in aree geografiche con costi della vita molto diversi, abbiamo purtroppo la negoziazione standardizzata e manca una vera negoziazione di area o di secondo livello.

stabilendo che nel privato tutto si può fare e nessuno interviene nel regolamentare quanto si deve retribuire una prestazione. Nel momento in cui, però, le aziende chiedono un aiuto di Stato, perché si trovano in grosse difficoltà, questo aiuto non deve finire in una ripartizione collettiva dello sforzo, cioè il denaro pubblico non può andare ad appannaggio di pochi manager

signor Ministro, la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese deve avvenire perseguendo l'obiettivo di realizzare una vera democrazia economica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 46 della nostra Costituzione. Per tali ragioni, non basta aprire ai lavoratori nuove prospettive di partecipazione diretta al capitale delle imprese; non basta assicurare la presenza dei rappresentanti dei lavoratori nei consigli di sorveglianza. Tutto questo non basta. In realtà, l'interesse dei lavoratori oggi non è quello di diventare dipendenti azionisti o di cogestire l'azienda in cui lavorano; ciò che interessa i cittadini in questo periodo di crisi è innanzitutto di essere lavoratori, avere un lavoro e, soprattutto, di disporre di una serie di strumenti che garantiscano la reale circolazione delle informazioni, nonché la conoscenza e il monitoraggio costante delle strategie societarie adottate e del livello di produttività conseguito. Solo in questo modo i lavoratori rafforzeranno concretamente le loro tutele. Solo in questo modo la gente potrà evitare di essere licenziata a sorpresa. Solo così i lavoratori parteciperanno, a pieno titolo, alla gestione della loro azienda e della loro vita senza avere bisogno di altro. Chiediamo, dunque, a nome dell'Italia dei Valori, cosa intenda fare al riguardo questo Governo, anche alla luce di quanto sta accadendo in FIAT e nella nuova FIAT-Chrysler-Opel. aprendo il XVI Congresso nazionale della CISL, il segretario generale Bonanni ha, tra l'altro, affrontato il tema della democrazia economica come risposta, possibile e in parte, alla crisi e al progressivo impoverimento delle pensioni e dei bassi salari. Devo dirle che noi siamo d'accordo con lui: pensioni e salari, soprattutto in questo momento di crisi, sono una vera e propria emergenza nazionale. Anche per questa ragione, vi è la necessità di una legge di attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, una legge che disciplini la partecipazione dei lavoratori alla *governance*, agli utili e all'azionariato collettivo. Tutto ciò, però, non basta; noi riteniamo vi sia anche la necessità di un nuovo patto tra capitale e lavoro, che affronti il nodo delle riforme strutturali, chieste dal Presidente di Confindustria anche da una parte del sindacato, riguardanti ovviamente le pensioni; una riforma integrale degli ammortizzatori sociali, con l'estensione delle garanzie ai lavoratori precari; una riforma dello Statuto dei lavoratori, nonché dell'efficacia e della struttura dei contratti collettivi. Ci interessa comprendere qual è al riguardo l'opinione del Governo.

quando si decise l'introduzione di una tassazione definitiva agevolata, nella misura del 10 per cento, per tutte le componenti della retribuzione collegate con indicatori di produttività o con gli utili dell'impresa. Intenzione del Governo era, cioè, sin da quel momento, di favorire quanto più possibile un cambiamento di quel modello di contrattazione collettiva, cui si deve la definizione dei salari nel nostro Paese, che fu definito nel 1993 in termini tali da aver generato, negli anni successivi, andamenti piatti (cioè, sostanzialmente uguali per tutti) e soprattutto moderati delle retribuzioni.

indicando un pericolo, quello dell'inflazione, che in realtà era appartenuto al decennio precedente e che era stato opportunamente contrastato con il cosiddetto accordo di San Valentino, allo scopo di un più generale controllo dei redditi, non solo di quelli di lavoro, ma anche, allora, delle tariffe dei prezzi amministrati, mentre, nel 1993, il problema non era più l'inflazione, come non lo sarebbe stato particolarmente negli anni successivi, ma la competitività. Pertanto, sarebbe stato già allora possibile fare quello che si è fatto ora, cioè collegare i salari con gli incrementi di produttività e - io aggiungo - con gli utili stessi dell'impresa, in modo che i salari possano crescere lì dove vi sono le condizioni obiettive perché crescano, ovviamente sulla base di una evoluzione solidale del salario, definita dalla contrattazione collettiva nazionale. questo è il nuovo modello contrattuale che è stato, su impulso dello stesso Governo che poi lo ha sottoscritto, realizzato da tutti gli attori sociali, con l'unica autoesclusione della CGIL, che appare ancora ancorata all'idea

il reddito viene definito sui vagoni più lenti del convoglio. È solo nella dimensione aziendale che quei redditi possono ulteriormente salire, tanto più se incoraggiati da una tassazione favorevole, favorevole, come quella che abbiamo introdotto fino a 35.000 euro e per 6.000 euro di componenti aggiuntive del reddito, tale da includere sostanzialmente tutti gli operai e gli impiegati. L'obiettivo è quello di di ampliare questa platea e di condurre a regime la disposizione che abbiamo introdotto. Peraltro, in questo tempo di crisi, abbiamo voluto proteggere diffusamente il reddito di coloro che sono costretti all'inattività dalla caduta della domanda globale, attraverso un programma straordinario di cosiddetti ammortizzatori sociali, rivolti, da una parte, soprattutto a mantenere vivo il rapporto di lavoro, in modo che il lavoratore resti occupabile, e, dall'altra, a far sì che l'azienda, la base produttiva del Paese, siano pronte a ripartire non appena le condizioni di ripresa si manifestino compiutamente in generale o per quel determinato segmento. Su tutto ciò si innesta il favore dichiarato di questo Governo per la partecipazione dei lavoratori, in primo luogo - lo sottolineo - agli utili dell'impresa, perchè questo deve essere lo scopo principale. Molti lavoratori, in questo tempo di crisi, ci hanno detto: quando le cose andavano bene non ce ne accorgevamo, il nostro salario rimaneva lo stesso, non subiva incrementi in relazione agli andamenti positivi dell'azienda, dei quali non partecipavamo; ora, invece, ci accorgiamo che le cose vanno male, perché siamo costretti al licenziamento o alla cassa integrazione. Ebbene, dobbiamo fare in modo che il lavoratore partecipi del rischio d'impresa anche

Le modalità possono essere diverse, si dovranno individuare liberamente e responsabilmente da parte degli attori sociali, azienda per azienda, e quindi è opportuno che il regolatore dia luogo ad un insieme di opportunità, che possono essere variamente scelte nelle diverse condizioni. Dico subito che consideriamo con una certa diffidenza il fatto che i lavoratori vengano chiamati a partecipare del capitale magari di una società prossima al fallimento. Quello forse è il momento meno idoneo per avviare esperienze di partecipazione dei lavoratori ai destini dell'impresa e probabilmente anche il momento più sospetto per un'invocazione di questo tipo. Invece, è proprio nella situazione situazione che vivono oggi molte imprese, di attesa di un tempo migliore ma di capacità positive dell'impresa stessa, che si possono realizzare quei patti chiari che danno luogo ad un'amicizia lunga tra le parti sociali, tra gli imprenditori e i lavoratori in una nuova fase di collaborazione che superi definitivamente il vecchio conflitto ideologizzato. Proprio in questo tempo, infatti, si condividono le fatiche per ripartire, ma è giusto che i lavoratori sappiano se potranno condividere anche gli esiti di quelle fatiche nel momento in cui le loro stesse fatiche daranno luogo a utili significativi per l'impresa. Seguiamo ovviamente con particolare attenzione il caso FIAT. La prossima settimana convocheremo le parti sociali perché cominciano a delinearsi elementi sufficienti sufficienti per iniziare un negoziato, un dialogo, al centro del quale poniamo la difesa dei siti produttivi italiani, perché vi sono ragioni oggettive per ritenere che questi siti possano essere performanti, anche nel contesto della riorganizzazione di un grande attore globale nella produzione di autovetture. Concludo con una considerazione rivolta al senatore Divina, a proposito della necessità e dell'opportunità, su cui questo Governo concorda, tanto che vi è già una proposta di legge del senatore Castro da noi condivisa, che vi debba essere un limite alle retribuzioni del *management* delle imprese quando queste o sono concessionarie di pubblici servizi o sono di proprietà pubblica o sono, in certa misura diretta o indiretta e nei limiti consentiti dall'Unione europea, sostenute da incentivi di carattere pubblico, proprio perché l'equa distribuzione della ricchezza significa non egualitarismo, ovviamente, non soluzioni uguali per tutti, ma soluzioni che siano percepite come eque in quanto correttamente ripartite tra tutti gli attori dell'impresa in proporzione al loro grado di responsabilità e al loro contributo ai risultati che l'impresa è in grado di generare.

tra garanzie e opportunità ci aiuterà a prevenire gli effetti più acuti di questa crisi e dei suoi inevitabili conflitti, ma soprattutto a costruire quella società attiva,

Presidente, prendo atto delle considerazioni che il Ministro ha svolto. Vedremo, nel percorso parlamentare del disegno di legge sulla partecipazione, se effettivamente le finalità da lui indicate saranno perseguite. Noi ribadiamo la volontà di puntare su una partecipazione scelta, in via contrattuale,

adottare soluzioni normative, sia pure d'iniziativa governativa, che prevedano di legare gli utili aziendali ai superstipendi dei manager, considerata la miriade di crack a cui abbiamo assistito nell'ultimo anno. Ciò di cui si deve occupare il Governo è tutelare i lavoratori, anello debole della catena produttiva, che devono sempre essere salvaguardati dalla condivisione dei rischi aziendali. Signor Presidente, signor Ministro, nonostante l'apprezzabile sforzo del suo lavoro, di cui bisogna darle atto, noi ci riteniamo insoddisfatti non per le cose che ha detto su alcune questioni poste nel corso del *question time*, ma sulla politica complessiva del Governo rispetto alla crisi. Infatti, il tema dell'attuazione dell'articolo 46 della Costituzione è collegato alla necessità e al nodo politico di affrontare una serie di riforme strutturali. Abbiamo la sensazione che stiate sprecando un'occasione importante, disponendo voi di un consenso politico e sociale molto ampio delle parti sociali e della vostra maggioranza politica per affrontare il nodo

Signor Presidente, al Ministro certo non sfugge, avendo lavorato egli stesso a lungo sui temi della sicurezza del lavoro, che è cresciuta una percezione, una salienza sociale, in ordine a questo tema. Vi sono ancora opinioni divergenti sul ruolo attivo delle parti sociali nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. quale ritiene il Governo possa e debba essere il compito svolto dagli enti bilaterali nella battaglia per un lavoro più sicuro, e con quali privilegiate articolazioni organizzative e funzionali si debba svolgere?

provocato dall'introduzione di alcune norme contenute nel suddetto decreto correttivo. Tale dibattito ha visto la partecipazione di importanti giuristi, i quali hanno paventato il rischio che tali norme possano modificare la giurisprudenza, attraverso un alleggerimento delle responsabilità penali, e che le stesse possano essere di nocumento ai processi in corso. In tale discussione sono intervenute associazioni di parenti delle vittime di incidenti sul lavoro, rappresentanze sindacali, forze politiche, nonché alte cariche istituzionali.

intende apportare, soprattutto come intende riformulare l'articolo 2-*bis*, cioè quelle parti del decreto che riguardano gli enti bilaterali che, in qualche modo, esautorano le Regioni e altri istituti pubblici, e

ha ribadito un consolidato orientamento giurisprudenziale che vuole che il datore di lavoro, in forza delle disposizioni specifiche previste dalla normativa antinfortunistica e di quella generale di cui all'articolo 2087 del codice civile, sia il garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale del lavoratore, con la conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo gli viene addebitato in forza del principio per cui non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo Signor Ministro, lei ricorderà certamente che, in una sua recente audizione presso la Commissione d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro, ebbi già modo di esprimerle, come giurista e come politico, tutte le mie perplessità sull'articolo 15-*bis* del decreto correttivo del decreto legislativo n. 81 del 2008. Ricordo che la lettera *d)* di questo articolo recita che il «non impedire l'evento equivale a cagionarlo» a condizione che «l'evento non sia imputabile» ad alcuni soggetti, fra cui - cito - capireparto, responsabili di stabilimento, ma soprattutto lavoratori.

rischieremmo di dare un colpo di spugna su alcuni processi pendenti e andremmo in una direzione antistorica rispetto agli orientamenti giurisprudenziali, non solo del nostro Paese, ma anche dell'Unione europea, considerata

lavoratori e delle imprese e della loro competitività, ma anche quello dei controlli e della prevenzione. Infatti, noi possiamo scrivere tutte le norme di questo mondo, anche le più belle, le più efficaci, le più europee, le più adeguate, ma se poi non abbiamo gli strumenti per controllare, dagli ispettori del lavoro alla ristrutturazione dell'Istituto che si deve occupare di questo settore, è chiaro che esse restano solo ed esclusivamente una voce nel deserto. Ci interessa comprendere quali strumenti per l'accertamento e la prevenzione

il Governo considera il diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro un diritto fondamentale, al quale si aggiungono ragionevolmente altri due diritti altrettanto fondamentali, quello al continuo incremento della conoscenza e della competenza per il lavoratore, in modo da essere sempre occupabile,

non è ancora efficacemente tutelato, perché, nonostante dal 1963, con una piccola eccezione nel 2006, i casi più gravi e mortali siano in costante diminuzione - considerando anche il fatto che più di metà degli infortuni mortali avviene sulla strada, perché riguardano persone che lavorano sulla via o che si spostano da casa al lavoro e viceversa - permangono significativi livelli di infortunio che devono essere ricondotti ad una dimensione molto, molto più contenuta e fisiologica.

soltanto di carattere formalistico e repressivo. Occorrono certamente regole, anche formali, occorrono sanzioni che le sostengano, ma c'è una soglia oltre la quale le regole formali e le sanzioni, soprattutto se esasperate, possono produrre l'effetto opposto, cioè allontanare la responsabilità dell'imprenditore

che, se applicati in misura fredda, possono nei fatti non generare quella effettiva sicurezza che poi determina la prevenzione di un infortunio, soprattutto di carattere grave o mortale. Per questa ragione abbiamo inteso promuovere un piano straordinario di investimenti nella formazione e nell'informazione, integrando le nostre risorse con quelle dei principali enti dedicati (INAIL e ISPESL) e con quelle di attori collettivi, come le rappresentanze

di tutte le organizzazioni imprenditoriali, comprese quelle vicine alla sinistra politica (penso alla contrarietà della Lega delle cooperative, della Confesercenti o della CNA, l'organizzazione di artigiani più vicina all'opposizione), abbiamo cercato, e continueremo a cercare, un'intesa più ampia che abbia quale scopo la collaborazione tra le parti sociali, la collaborazione che si realizza attraverso enti bilaterali e comitati paritetici. Non credo che si possa rinunciare a queste soluzioni, senatore Nerozzi, perché sono il contenuto di intese intervenute con CISL, UIL, UGL e con tutte le organizzazioni dei datori di lavoro, quindi, con un consenso molto molto ampio (che purtroppo non vede d'accordo la CGIL) di tutte le altre organizzazioni circa la valorizzazione delle forme cooperative fra le parti sociali per investire adeguatamente nella sicurezza. Circa, infine, la norma la norma citata da molti interroganti, voglio ricordare che ha un solo scopo: quello di precisare gli ambiti della responsabilità del datore di lavoro, che non è il manager lontano, ma è l'artigiano, il commerciante, il coltivatore diretto. qual è l'ambito della sua responsabilità quando appare prevalente, se non addirittura esclusiva, la responsabilità di uno dei sottoposti della lunga filiera? noi dobbiamo certamente mantenere la responsabilità del datore di lavoro nel vigilare a che siano state approntate tutte le condizioni di sicurezza nel lavoro, ma allo stesso tempo ‑ credo che lei ne

testo proposto può non essere quello più idoneo, può dare luogo a fraintendimenti. Io non credo, ma poiché ci sono dubbi in proposito, noi abbiamo detto che lo cambieremo: non che siamo disponibili a cambiarlo, ma che lo cambieremo. E lo faremo nel momento in cui dovremo e potremo farlo, cioè dopo i pareri delle Commissioni parlamentari e l'ulteriore dialogo con gli attori sociali, nel momento in cui, in seconda lettura, il Consiglio dei ministri darà il via definitivo al decreto delegato correttivo, nell'ambito dei principi e dei criteri della legge varata dalla maggioranza di allora e dal Governo Prodi nella scorsa legislatura.

della responsabilità del datore di lavoro e di tutti gli attori che compongono quel livello di sicurezza e di flessibilità che sotto la parola *flexsecurity* trova la sua sintesi.

*(IdV)*. Io ringrazio il Ministro e prendo atto delle buone intenzioni. Il Gruppo dell'Italia dei Valori si dichiara fin da ora disponibile a dare dare suggerimenti e ad aiutare a meglio riformulare quell'articolo e, soprattutto, ad intervenire su quell'attività di prevenzione e formazione che il Ministro ha ricordato

Signor Presidente, noi riteniamo che sia stata opportuna la precisazione del signor Ministro con riferimento all'ambito e ai confini entro cui si muovono i decreti correttivi del Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Dobbiamo però comprendere che se si vuole introdurre un diritto penale speciale riguardante questa materia, certamente la sede non può e non deve essere solo ed esclusivamente quella legata

si avvale per i controlli e la prevenzione sia insufficiente. Su questo tema dobbiamo investire molto di più perché servono più ispettori e più gente che controlla, anziché più norme di difficile applicazione. Fino a quando non perseguiremo e raggiungeremo questo obiettivo, possiamo fare tutte le disquisizioni

del Governo, colleghi, l'Italia spende meno della metà della media europea per le famiglie, e per questo è il Paese dove nascono meno bambini, dove ci sono pochi nidi e pochi servizi per i disabili e gli anziani. È il Paese che cresce meno, con l'occupazione femminile più bassa, ed è un Paese tra i più diseguali nel mondo occidentale. Occorre una svolta: più risorse e servizi alle famiglie, in particolare da quelle con figli, a partire dal primo, con disabili e anziani non autosufficienti. Il Governo, all'opposto, ha abolito il Ministero della famiglia e ha tagliato tutti i fondi per la famiglia. La riduzione prevista per il 2009 è pari a meno 21,8 per cento e arriverà a meno 55,9 (pari a 1.777,5 milioni di euro) nel 2011. Dal 2010, poi, non sono più previste risorse per i congedi parentali e per la non autosufficienza. Non crede il Governo che occorra aumentare del 35 per cento gli assegni familiari, a partire dal primo figlio, estendendoli anche agli autonomi? E non crede che si debba subito stanziare un miliardo di euro per i nidi e i servizi agli anziani? E non è necessaria la gratuità dei libri di testo? Inoltre, per chi perde il posto di lavoro, non è urgente un sostegno per la retta dei nidi e sgravi per i carichi familiari e per l'educazione dei figli? La famiglia non può essere lasciata sola, specialmente nella crisi; non è un costo, è il miglior investimento per uscire dalla crisi.

non sono stati di carattere strutturale, ma solo di carattere monetario e *una* *tantum*. Ne sono esempi lampanti il *bonus* famiglia, la *social* *card* e il fondo di credito per i nuovi nati. Nulla però è stato fatto per favorire una maggiore conciliazione tra lavoro e famiglia. Addirittura, sono state varate politiche che hanno reso più difficile la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, come i tagli all'organico del corpo docente e la detassazione degli straordinari; una misura - come è noto - che può essere applicata solo nei confronti dei lavoratori che fanno o possono fare gli straordinari, quindi i soli uomini, signor Ministro, dato che non credo che le donne con figli piccoli possano farli. Queste scelte hanno provocato l'effetto di bloccare il tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro, che quest'anno non è aumentato neanche di un punto percentuale. Per tali ragioni chiediamo quali provvedimenti intenda assumere l'attuale Esecutivo al riguardo, garantendo al contempo l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze di genere nel mondo del lavoro. Presidente, l'ISTAT afferma che per l'anno 2007 sono 2.635.000 le famiglie che si aggirano o stanno al di sotto della cosiddetta soglia di povertà, pari all'11,1 per cento delle famiglie residenti italiane. Il termine povertà non viene usato, ma oggi è purtroppo drammaticamente di attualità, se consideriamo che vi sono 7.542.000 italiani che vivono al di sotto della soglia di povertà, e sono circa il 12,8 per cento della popolazione italiana. Un altro dato drammatico e sconfortante, diramato dall'ISTAT, è che il 3,7 per cento delle famiglie ha un livello di spesa solo di poco superiore alla soglia di povertà. In poche parole, la crisi strutturale e quella congiunturale rendono le famiglie italiane meno ricche e più indebitate. Nonostante ciò, le famiglie italiane rappresentano il più grande ed efficace ammortizzatore sociale e per questo i figli oggi si rifugiano ancor di più, in età avanzata, all'interno della famiglia stessa. I rimedi che il Governo in questo anno ha proposto riguardano il *bonus* famiglia, che da un suo primo esame risulta parzialmente adeguato ai bisogni, e la *social card*. Noi riteniamo che vi sia bisogno di maggiori interventi e comunque di interventi che siano più generali, soprattutto in questo momento di crisi particolare, e che sia necessario concentrare le risorse investendo sulla famiglia, anziché disperderle in mille rivoli che poi non producono gli effetti sperati. Vorremmo conoscere al riguardo l'opinione del Governo.

il Consiglio dei ministri ha varato nei giorni scorsi, con atto quindi collegiale, il Libro bianco sul futuro del modello sociale in Italia assunto a riferimento i valori codificati nella nostra Carta costituzionale, che sono stati riletti soprattutto in funzione della centralità della persona in sé, anche nelle sue prime proiezioni relazionali, come la famiglia e la comunità. La famiglia è quindi al centro dell'attenzione della politica di Governo. Essa certamente svolge la funzione solidale che le è riconosciuta anche in questo tempo di crisi, oltre ad essere la cellula vitale che consente la riproduzione della della nostra società, ed è per questo che la famiglia, intesa come unione tra un uomo e una donna, meglio se sostenuta da un vincolo matrimoniale e votata alla procreazione, costituisce il il rapporto affettivo che presenta un interesse pubblicistico, da non confondere con altri rapporti affettivi che non hanno altrettanta valenza pubblica con conseguenti iniziative di sostegno. Noi pensiamo che sia necessario promuovere la famiglia e la sua diffusione, che sia necessario sostenere anzitutto l'anticipo nelle scelte responsabili di vita dei dei più giovani, perché molto spesso scuola, lavoro, matrimonio, natalità (a quel punto davvero difficile) tendono a spostarsi troppo in avanti e dobbiamo invece garantirne un adeguato anticipo, quanto meno come accade in molti altri Paesi, evitando quello che il senatore Livi Bacci chiama opportunamente "fenomeno dei giovani vecchi". Noi dobbiamo sostenere la conciliazione fra tempo di vita e tempo di famiglia dei coniugi che lavorano, e a ciò devono soccorrere modelli di contrattazione collettiva che consentano di modulare l'orario di lavoro, senso stiamo sollecitando le parti sociali. Allo stesso modo, occorre una maggiore diffusione dei servizi di cura all'infanzia, che non si risolve soltanto nelle tradizionali strutture pubbliche o private, anche aziendali o interaziendali, ma anche nella diffusione di servizi a cura di famiglie, nell'ambito di regolazioni di tipo regionale, che intendiamo favorire attraverso un modo semplice di remunerare queste attività di cura

allora tutto il nostro impegno per costringere entro limiti certi di finanza pubblica i servizi socio-sanitari del Centro-Sud del Paese, che non erogano adeguati servizi alla non autosufficienza, perché i loro modelli organizzativi sono assolutamente obsoleti e fondati solo sulla spedalità, della rimanente area del Centro che funziona e del Nord, dove troviamo un adeguato spazio ai servizi territoriali, tra i quali quelli assistenziali che si integrano con quelli socio-sanitari, e che sono dedicati soprattutto soprattutto alla non autosufficienza. Il reddito è stato sostenuto certamente anche con misure immediate, come ci consigliano i documenti internazionali, che dicono ai Governi di adottare misure mirate, tempestive

un intervento su quel terzo di famiglie che possiamo ritenere più disagiate con il cosiddetto*bonus* famiglia, quella sorta di quattordicesima rivolta ai lavoratori dipendenti, in relazione al loro contesto familiare, da un minimo di 200 a un massimo di 1.000 euro; abbiamo sostenuto i mutui per l'acquisto della prima casa; abbiamo diffuso tariffe agevolate per l'utenza domestica di elettricità e di gas;

di famiglie del bisogno assoluto - o perché caratterizzate da persone anziane o perché vi sono minori in contesti familiari di povertà assoluta alle quali vengono trasmessi i primi aiuti attraverso questa sorta di infrastruttura costituita dalla carta elettronica anonima, che potrà essere domani il veicolo per molte altre provvidenze. un lato, dall'individuazione di una prima platea del bisogno assoluto, che dovrà essere ulteriormente affinata (basti pensare alla necessità di correggere e adattare l'indicatore relativo alla situazione il canale di comunicazione rappresentato della carta di credito si realizza oggi, ma per durare e per essere funzionale alla trasmissione di ben altri aiuti. Insomma, molti sono stati gli interventi, ma l'appuntamento principale che dovremo affrontare in questa legislatura sarà il passaggio, o meglio

in modo da abbattere il reddito in rapporto ai carichi di famiglia, così che la tassazione successiva degli enti locali si realizzasse sul reddito reso netto dai carichi di famiglia. Il Governo successivo, invece, con il ministro Visco, ha sostituito le deduzioni con le detrazioni, che hanno ridotto la tassazione centrale per i carichi di famiglia, mantenendo però inalterato il reddito lordo, così che la tassazione locale è poi intervenuta pesantemente e in maniera punitiva nei confronti delle famiglie più numerose. Il nostro obiettivo, ovviamente, considerando le condizioni di finanza pubblica che si potranno determinare nel momento della ripresa, è di tornare all'idea (che era nostra e che come tale ribadiamo) di abbattere il reddito in relazione ai carichi di famiglia, riconoscendo così il fisco l'importanza del nucleo familiare più numeroso.

affermato che il*bonus* fiscale di Tremonti e Sacconi per l'82 per cento non va a famiglie con figli e per questo è una scelta "che va contro la famiglia".

tutti gli indicatori dell'ISTAT. Se il Governo vuole fare qualcosa intanto aumenti gli assegni familiari, iscriva - come noi chiediamo - all'ordine del giorno le leggi sui nidi e sulla non autosufficienza, che sono d'iniziativa popolare, e soprattutto non tagli i fondi ma li ripristini. Altrimenti, non avremo politiche

Ne ha facoltà. CARLINO *(IdV)*. Signor Ministro, la ringrazio per la risposta, che tuttavia mi lascia insoddisfatta. Mi preme ricordare che sul tema della conciliazione lavoro-famiglia, durante la scorsa legislatura, con la finanziaria del 2007, sono stati previsti vari interventi a sostegno della maternità e della paternità, soprattutto per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, come, ad esempio, l'estensione della possibilità di usufruire del congedo parentale

si traducano in fatti concreti. Inoltre, signor Ministro, vorrei dirle che con le "umilia *card*", come noi dell'Italia dei Valori le abbiamo ribattezzate, non si possono davvero risolvere i tanti problemi delle famiglie italiane. Signor Ministro, noi siamo ovviamente interessati a confrontarci con il Governo e particolarmente con lei sui temi e sulle questioni poste dal Libro bianco. Dobbiamo però prendere atto, con profondo rammarico, che il Governo e la maggioranza avevano promesso il quoziente familiare come strumento di riequilibrio sociale e che questo è stato definitivamente abbandonato, e che, degli unici due strumenti messi in campo, la *social card* appare inadeguata per le difficoltà di accesso e per i limiti di reddito (pare costi di più di quanto valga) e, come è stato già ricordato, il *bonus* famiglia, oltre ad essere una misura *una tantum,* non interessa prevalentemente le famiglie con figli, anzi, produce anche effetti distorti in caso di convivenze, perché è previsto che si raddoppi il *bonus*. Ora, rispetto a questo, io credo che una politica accurata avrebbe dovuto concentrare le risorse solo ed esclusivamente sulle famiglie, in particolare sulle famiglie monoreddito, evitando di sprecare soldi nell'operazione Alitalia, vincolando di più le banche nelle modalità di concessione del credito alle famiglie ed incentivando le famiglie con figli (prevedendo, ad esempio, un contributo di 100 euro al mese per il primo figlio e di 50 per il secondo figlio per quelle famiglie che hanno un reddito familiare fino a 50.000 euro). Per queste ragioni riteniamo insoddisfacente la sua risposta.